molto brevemente. Esattamente 38 anni fa, alla stessa ora in cui oggi iniziano i nostri lavori, in Piazza Fontana, a Milano, esplodeva una bomba presso la Banca dell'agricoltura. 13 persone morirono sul colpo, altre 3 morirono successivamente per le ferite riportate ed 80 furono coloro che rimasero segnati permanentemente da quell'evento. Cominciava così quella che Sergio Zavoli, che oggi siede con noi in quest'Aula, definì una "lunga notte della Repubblica". Sulla dialettica democratica, sulla politica delle idee e dei movimenti, sul dispiegarsi delle lotte sociali e sindacali di quegli anni si allungava l'ombra di intrighi e di trame feroci. A quei primi morti, tanti altri se ne aggiunsero per gli attentati al treno "Italicus", a Brescia, a Bologna, nella follia delle stragi fasciste e degli assassinii politici. Ma quella data rimane simbolica, perché segna l'avvio di un tentativo sciagurato di deviare il corso della democrazia attraverso l'intreccio di responsabilità individuali, di connivenze, di deviazioni di apparati dello Stato, di depistaggi. Un tentativo cui si oppose una forte richiesta di verità e di giustizia che ha unito coloro che erano stati colpiti nella loro carne e nei loro affetti alla battaglia civile per il riscatto della nostra democrazia. Una battaglia che ha segnato, signor Presidente, un'intera generazione. Un desiderio di verità e di giustizia che è ancora inappagato e che si ripropone di fronte ad eventi più recenti. Il ricordo di quelle vittime non può fermarsi alla sola e necessaria solidarietà umana, che tutti naturalmente condividiamo, ma richiede a noi stessi l'impegno concreto di non ignorare quel bisogno, di non smettere di trovare la via con tutti i mezzi che ci mette a disposizione la nostra Costituzione, per recidere ogni legame sotterraneo, ogni omertà, ogni copertura, ogni tentativo di aggiustare la verità su quegli eventi e su quelli più recenti, a cominciare da quell'altra notte della Repubblica, che a Genova ha prodotto una tragica sospensione della democrazia (mi avvio a concludere, signor Presidente) in piazza Alimonda, alla scuola Diaz e Lo dobbiamo a tutte le vittime, a noi stessi e a questo Paese e alle nostre istituzioni democratiche. Per questo, la data del 12 dicembre 1969, sebbene lontana nel tempo, non può richiamarci al solo dovere del ricordo, ma rappresenta ancora oggi un evento di bruciante attualità.

Comunico che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi a conclusione della seduta antimeridiana, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 19 dicembre. L'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi prevede la discussione dei disegni di legge in materia di semplificazione di adempimenti amministrativi sanitari, contributo allo *Staff College* ONU di Torino e contributo alla sede italiana della Delegazione palestinese. Sempre oggi pomeriggio, alle ore 18, avrà luogo l'informativa urgente del Vice Ministro agli affari esteri sui recenti attentati in Algeria. I Gruppi potranno intervenire per 10 minuti ciascuno (15 minuti al Gruppo misto). Pertanto la seduta potrà proseguire anche oltre le ore 20. Resta confermato che nelle due sedute di domani si svolgerà la discussione generale sul disegno di legge collegato relativo al protocollo su lavoro e previdenza, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. La Presidenza ha inoltre avuto mandato dalla Conferenza dei Capigruppo, tenuto anche conto dell'andamento delle trattative con i rappresentanti degli autotrasportatori, di intraprendere contatti con il Governo al fine di prevedere un'eventuale informativa del Ministro dei trasporti domani pomeriggio alle ore 18, cui potranno seguire gli interventi dei Gruppi con le modalità

si è intanto stabilito che l'Assemblea non terrà seduta nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 dicembre, che saranno pertanto riservate ai lavori della 5a Commissione permanente e delle altre Commissioni competenti in sede consultiva. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 19 dicembre, con due sedute alle ore 9,30 e alle ore 16, per la discussione generale congiunta dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella giornata di martedì 18 dicembre per definire l'organizzazione dei lavori dei successivi giorni della settimana, relativamente ai documenti finanziari e al seguito della discussione del Protocollo su lavoro e previdenza. Non appena trasmessi dalla Camera dei deputati i disegni di legge finanziaria e di bilancio saranno immediatamente deferiti alla 5a Commissione permanente. Salvo i diversi termini che potrebbero essere comunicati in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati, le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione bilancio entro le ore 13 di martedì 18 dicembre; la 5a Commissione permanente - come sopra ricordato - riferirà all'Assemblea a partire dalle ore 9,30 di mercoledì 19 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati entro le ore 18 di martedì 18 dicembre, salvo diverse determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

ho gia detto, salvo diversi termini che potrebbero essere comunicati in relazione ai tempi di trasmissione della Camera dei deputati, le Commissioni permanenti dovranno presentare i rapporti alla Commissione bilancio entro le ore 13 di martedì 18 dicembre. Gli emendamenti

dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea

nulla. Abbiamo necessità di sapere quando lavorare sugli emendamenti per la Commissione prima di questa comunicazione, perché altrimenti crediamo che martedì si possono presentare, mentre in realtà non è così. Appena arriveranno i provvedimenti finanziari - così gli Uffici mi stanno riferendo - i Presidenti delle Commissioni comunicheranno ai Presidenti dei Gruppi i termini per la presentazione degli emendamenti,

cercheremo di definire un programma dei lavori della Commissione che sia compatibile con la decisione, che anche io - come tutti gli altri senatori - apprendo ora, di fissare l'inizio dei lavori dell'Aula sui disegni di legge finanziaria e bilancio nella giornata di mercoledì. Quindi prevedo - lo dico ai colleghi senatori - che dovremo cominciare i lavori della Commissione, sulla base delle decisioni che comunque prenderemo assieme nell'Ufficio di Presidenza (non le prendo io da solo), già nella giornata di lunedì per esaminare i disegni di legge e già nell'Ufficio di Presidenza di domani definiremo comunque una scadenza per la presentazione degli emendamenti in Commissione che sia coerente con la scadenza della presentazione degli emendamenti per l'Aula,

che non sia presentato in Commissione non è presentabile in Aula. Quindi, certamente nell'Ufficio di Presidenza di domani fisseremo un termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione che sia compatibile con quello determinato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo per la presentazione degli emendamenti in Aula. Insomma, cercheremo di organizzare i lavori della Commissione in modo tale da risultare compatibili nella tempistica con gli obblighi e con le previsioni regolamentari e con il fatto che comunque bisogna garantire che la Commissione bilancio e le Commissioni di merito abbiano il tempo necessario per pronunciarsi, sia pure

il momento esatto nel quale la Camera dei deputati ci trasmetterà i due disegni di legge. Se lo conoscessimo con assoluta precisione, naturalmente potremmo essere già adesso di fissare scadenze che non sono ad oggi prevedibili, ma io spero che nella giornata di domani queste previsioni si possano fare.

mi consenta di sottolineare all'Assemblea la situazione che si è determinata in relazione all'esame del provvedimento collegato ai documenti di bilancio e al disegno di legge di riforma del sistema previdenziale del mercato del lavoro. Domani l'Assemblea ne inizierà l'esame

presentatori della gran parte degli emendamenti all'esame della Commissione e probabilmente anche dell'Assemblea, hanno riconosciuto che solo il voto di fiducia potrà consentire l'approvazione del provvedimento. Francamente, nella mia non breve esperienza parlamentare, non ho mai visto una maggioranza ricorrere all'ostruzionismo fin dal primo momento dell'esame di un provvedimento e lungo tutto il suo *iter*

Signor Presidente, signor Ministro,illustri colleghi, credo che il provvedimento che ci accingiamo a votare, probabilmente senza clamore, abbia invece un grande significato per i cittadini perché li aiuta nella loro vita quotidiana con molte semplificazioni nell'ambito sanitario e con alcune norme migliorative riferite all'assistenza sanitaria, specialmente nell'ambito della terapia del dolore.

contemplino la semplificazione attraverso l'abolizione di certificazioni oramai obsolete e superate dalle conoscenze scientifiche, dal miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e da altre strutture che oggi hanno preso il posto di precedenti controlli. Sono circa 20 le certificazioni che verranno abolite. In particolare, ricordo il certificato, di antica memoria, di sana e robusta costituzione, che veniva richiesto per tantissime situazioni, in maniera anche abbastanza illogica, come ad esempio per l'attività sportiva non agonistica o per svolgere l'attività di farmacista o ancora per alcuni posizioni del pubblico impiego e addirittura per la cessione del quinto dello stipendio;

altresì rivisto il concetto della certificazione di esonero dalle lezioni di educazione fisica: non si tratta più un fenomeno di tutto o nulla, ma della possibilità di certificazione e di accordo (tra il medico curante, la struttura ed eventualmente il medico della ASL) circa percorsi di motricità adatti anche a situazioni di *handicap* o, comunque, a difficoltà di carattere fisico. Inoltre, proponiamo l'abolizione delle certificazioni per partecipare a vacanze di carattere collettivo. Gli articoli 3 e 4 prevedono l'abolizione dei libretti sanitari e di altre certificazioni per le imprese alimentari, perché i controlli su questi settori sono oramai decisamente migliori attraverso altre disposizioni. Gli articoli 5 e 6 rinviano ad intese Stato-Regioni due argomenti importanti: da un lato, si prevede la possibilità di ricercare e

l'articolo 7 è importante e prevede la possibilità per Regioni e Province autonome di istituire registri che riguardino malattie d'interesse nazionale; si fa soprattutto riferimento ai registri tumori, che oggi non sono diffusi su tutto il territorio, o ad altre malattie quali l'AIDS, o ancora a registri per le cause di morte e per i portatori di protesi impiantabili (un settore che registra evidentemente un grande sviluppo e di cui mancano i dati epidemiologici).

L'articolo 8 tratta norme semplificative sull'uso degli stupefacenti. Credo che sia a tutti noto, signor Presidente, come il nostro Paese sia fortemente arretrato rispetto all'utilizzo di tali sostanze, probabilmente per ragioni di carattere culturale, ma anche per vincoli di carattere normativo. La norma prevede di semplificare la prescrizione di questi farmaci, che non dovrà più essere fatta in triplice copia su un prontuario particolare, ma su quello semplice regionale con cui si prescrivono tutti gli altri farmaci. Viene altresì semplificata la tenuta dei registri presso le strutture del Servizio sanitario per l'annotazione dell'uso di tali farmaci, ma soprattutto si introduce il concetto che questi farmaci possano essere utilizzati per il dolore severo di qualunque natura, che viene quindi considerato come sintomo e malattia da trattare di per sé, e non soltanto per il dolore severo legato a malattie di carattere neoplastico o degenerativo, come era precedentemente

così come la terapia domiciliare di pazienti in terapia sostitutiva con metadone o similari. Abbiamo inoltre previsto all'articolo 9 la confisca dei beni strumentali in caso di esercizio abusivo della professione medica per cercare di scoraggiare ulteriormente tale pratica abusiva.

era abolita. L'articolo 11 introduce la possibilità per le scuole di specializzazione, in accordo con le Regioni, di introdurre percorsi di subspecialità di durata non superiore a due anni, in maniera da poter avere percorsi diversificati all'interno delle scuole di specializzazione per sottospecialità oggi ormai presenti anche negli ospedali e nel Servizio sanitario. Completano la legge gli articoli 12 e 13, che conferiscono obbligo alle Regioni e alle Province autonome di completare la rete delle farmacie e anche di bandire un concorso straordinario per soli titoli per farmacisti, con norme che favoriscono l'impiego di giovani farmacisti sotto l'età di 40 anni. Sottolineo il fatto che, da più di dieci anni, i concorsi per le farmacie sono bloccati,

abbiamo presentato una serie di emendamenti sull'utilizzo degli alcolici nei pubblici esercizi. In particolare, crediamo vi siano emendamenti di buonsenso,

previsione che dopo le ore 2 nei locali nei quali si accede solo con l'acquisto di un biglietto d'ingresso la consumazione, eventualmente compresa, debba essere analcolica;

provvedimenti; programmi per incentivare il trasporto notturno dei giovani con mezzi pubblici e per l'accompagnamento a domicilio di chi non è in grado di mettersi al volante; l'estensione - come abbiamo detto - tutela dalla vendita alla fascia da 16 a 18 anni (cioè che non si possano più vendere alcolici ai minori di 18 anni); il divieto di vendita di alcolici in forma ambulante e che la loro somministrazione ed il loro consumo possano essere effettuati esclusivamente nei pubblici esercizi, evitando che esercizi commerciali e artigiani, focalizzati sulla somministrazione non assistita di alimenti e bevande e non soggetti alla specifica autorizzazione di pubblica sicurezza, divengano luoghi di consumo incontrollato. tutta un'altra serie di misure, compreso il divieto del cosiddetto *after hour* nel quale si spinge il pubblico a consumare alcolici riducendone il prezzo,

a quello delle bevande alcoliche; e infine, riguardo alle sanzioni per la mancata esposizione delle tabelle previste, prevediamo la sostituzione della sanzione della chiusura del locale con sanzioni di tipo pecuniario. A nostro avviso,

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1249, avente per oggetto «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute», non rappresenta un mero condensato di semplificazioni di alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle autorizzazioni sanitarie: è qualcosa, a nostro dire, di ben più complesso. Tale provvedimento piomba all'esame di quest'Aula, diciamocelo chiaramente, in un clima la cui attenzione è pari a quella che solitamente viene riservata alle mosse semplici, non strategiche e tanto meno fondamentali, che sono destinate soltanto a prendere tempo in quella più complessa partita a scacchi, che si disputa dentro e fuori dal Parlamento e che risponde al nome di finanziaria e di legge elettorale. Ma la riflessione, che pure dovrebbe svilupparsi sul presente disegno di legge, non può prescindere dall'interrogativo che si pone nei riguardi dell'opportunità di un'eccessiva semplificazione di questioni e problemi differenti, per i quali forse era preferibile usare una maggiore prudenza. Esiste il convincimento diffuso, nella pubblica opinione, che il nostro Paese sia stretto eccessivamente da un intenso groviglio di leggi che ne appesantiscono la funzionalità. Anche l'efficienza del Servizio sanitario nazionale è spesso compromessa dall'eccessiva incidenza di procedure burocratiche e, dunque, un provvedimento che nelle sue finalità è destinato ad agire in modo significativo e concreto sulla rimozione di procedure obsolete che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, come pure sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte, va condiviso. Ma (ed esistono fondate ragioni per alzare l'asticella del «ma») a condizione che venga sempre garantito e tutelato il diritto alla salute dei cittadini. Si rilevano, nell'articolato del presente disegno di legge, ragionevoli soppressioni di una serie di certificazioni che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, sembrano non avere più fondate ragioni per continuare ad esistere. Riteniamo ci sia poco da argomentare sull'eliminazione del certificato di sana e robusta costituzione fisica richiesto per l'iscrizione agli istituti magistrali e ai corsi per infermieri, corsi per infermieri, o del certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti; o del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego; o del certificato di idoneità psicofisica per l'attività di maestro di sci. Ma ci sia consentito rilevare che forse non è perfettamente sovrapponibile il confronto delle eliminazioni, cui sopra ho accennato, con l'abrogazione del certificato di idoneità fisica e psichica per svolgere l'attività di giudice onorario o di pace. Stante le finalità del presente disegno di legge, non riteniamo che possa essere considerata una disposizione, diretta a mettere un freno al fenomeno dell'abusivismo della professione sanitaria, la soppressione, prevista al comma 10 dell'articolo 1, riguardante le certificazioni relative all'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomelitica e contro l'epatite virale B, di cui all'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. La previsione dell'autocertificazione, così com'era contemplata nella stesura originaria del presente disegno di legge, in luogo dell'attuale obbligo di certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni sopra richiamate, non rappresenta una misura di garanzia necessaria e dunque sufficiente. La profilassi obbligatoria delle vaccinazioni realizzata nel nostro Paese ha consentito che alcune malattie, quali quelle sopra citate, siano state in questi anni definitivamente debellate. È però con una certa preoccupazione che dobbiamo registrare un preoccupante riesplodere, in coincidenza di un più marcato fenomeno immigratorio, di casi, ad esempio, di TBC, registratisi nelle scuole italiane, che sono espressione, appunto diretta dei prodotti di una società multirazziale con i quali necessariamente dobbiamo fare i conti. Non è discriminante, dunque, prevedere e modulare opportune politiche di prevenzione sanitaria, perché sarebbe invece un atteggiamento irresponsabile, e lo sarebbe ancor di più per il legislatore, non tenere conto delle mutate caratteristiche e delle trasformazioni socio-culturali avvenute nel nostro Paese. L'autocertificazione - ripeto - così com'era prevista nella stesura originaria di questo disegno di legge, a fronte anche di diverse sensibilità culturali e dunque sanitarie, non poteva e non può essere considerata una misura sufficiente di garanzia per tutti; e forse non è sufficiente nemmeno la trasmissione da parte dei dirigenti scolastici, come invece viene previsto nell'attuale redazione dell'articolo, degli elenchi degli alunni che vengono iscritti per la prima volta alla prima classe della scuola primaria, al competente servizio dell'azienda sanitaria locale, ai fini della conoscenza dell'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie. La semplificazione non può essere sinonimo di un imbarazzante semplicismo che rischia di compromettere la sicurezza, il diritto alla salute che deve invece essere garantito verso tutti e soprattutto, nei confronti dei bambini che accedono alla scuola dell'obbligo. Lo stesso ragionamento che sin qui abbiamo sviluppato, riteniamo necessario estenderlo anche a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 dello stesso disegno di legge, riguardante l'eliminazione di presentazione del certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori. L'interrogativo di fondo che dunque ci poniamo è: occorre considerare prioritaria l'eliminazione di un procedimento che, stante i ritmi della società moderna, può persino apparire come un'inutile perdita di tempo, occorre indurre, anche sotto il profilo della pur antipatica (lo riconosco) rigidità procedurale, al rispetto di norme attestanti maggiori garanzie per tutti? Io opterei per la seconda scelta. L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), abroga gli obblighi relativi al libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione degli alimenti; lettera *b)*, sopprime l'obbligatorietà del certificato medico che esclude il pericolo di contagio, ai fini della riammissione al lavoro degli alimentaristi summenzionati dopo un'assenza di durata superiore ai cinque giorni per malattia. Ora, anche qui, trattandosi di norme che incidono sulla sicurezza alimentare, riteniamo opportuno non farci travolgere dal «costi quel che costi» che nasce dalla smania di semplificazione eccessiva. Noi riteniamo di poter convergere verso la definizione di un giudizio positivo sul presente disegno di legge, in quanto riteniamo che l'obiettivo principale, quello cioè riguardante in ogni caso «il continuare a realizzare ed assicurare la tutela della salute pubblica», non sia stato affatto conseguito. A nostro giudizio, sono stati mescolati in questo disegno di legge troppi ingredienti. troviamo: la sana e robusta costituzione fisica; i difetti dei farmacisti che partecipano ai concorsi; l'idoneità fisica dei responsabili tecnici per i servizi di autoriparazione; la tessera sanitaria per gli addetti ai lavori domestici; il divieto di vendita e somministrazione di alcolici negli autogrill autogrill autostradali; la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria; la semplificazione dei vari registri da parte dei farmacisti per il controllo del movimento degli stupefacenti; i farmaci per il trattamento del del dolore severo; le disposizioni in materia di polizia mortuaria. La sensazione, di fronte a questa miscellanea di ingredienti, è quella di avere a che fare con un sorta di maionese impazzita. Quindi, prima di raggiungere di raggiungere questo non auspicabile risultato, invitiamo il Senato, quest'Assemblea, a valutare il provvedimento con serietà e ad usare qualche cautela in più.

garantito. La presenza del Ministro mi dà la possibilità di rivolgere un appello

a livello nazionale e dopo le vicende di ieri della Calabria, non è facile immaginare che una Regione venga commissariata perché è scattato il sistema sanitario di emergenza. Questo è quindi un principio importante, un principio forte a cui il Governo ha voluto ricorrere.

merito alla formazione, si può porre il problema di creare 20 o 21 sistemi di formazione a livello nazionale. Mi auguro, quindi, che l'Agenzia nazionale - sono sempre più favorevole a rafforzare

eticamente scorretto immaginare che c'è chi nasce fortunato perché nasce in una Regione e chi nasce sfortunato perché nasce in un'altra Regione; quindi, anche sul tema di formazione abbiamo inserito un richiamo, e rivolgo un appello al Ministro perché so che in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà scendere nel particolare.

a Commissione igiene e sanità e Commissione industria. Quindi, è un tema di attualità. Su questo argomento penso che la formulazione del testo ora al nostro esame ci possa in qualche modo dare soddisfazione, ma soprattutto ci può dare soddisfazione il fatto che da questo ci è consentito avanzare

di fronte ad un disegno di legge che si pone come obiettivo una semplificazione che va a favore di tutti i cittadini, è chiaro ed evidente che ci si deve schierare aderendo favorevolmente nel tentativo di fare il meglio, cosa che noi abbiamo fatto in maniera positiva fin dall'inizio. Va ricordato che verso quest'obiettivo il testo originale si presentava con un regolatorio molto confuso, spesso ignaro delle determinazioni già acquisite da alcune Regioni e, come ha ricordato la collega Monacelli, con una pletora di argomenti. Tuttavia, il lavoro è stato costruttivo e proficuo, e così si è trovata una migliore omogeneizzazione sulle vaccinazioni, sulle disposizioni alimentari, soprattutto sui registri delle patologie, dei farmaci *off label* e sul regolatorio delle farmacie. Credo sia assolutamente ingiusto e non corretto attribuirsi diverse penne del pavone per questi miglioramenti, perché lo ha stabilito la Commissione al suo interno, nel suo insieme, e credo sia un fatto estremamente positivo.

e, soprattutto, ad altri tavoli si sta discutendo delle medesime argomentazioni. Condivido quindi quello che ha ricordato il senatore Cursi a proposito delle farmacie e mi unisco anch'io alla pressante richiesta al Presidente del Senato

In ogni caso, altri confronti ci potranno aspettare su questi temi, così come possibili ulteriori miglioramenti possono venire dagli emendamenti presentati in Aula.

Presidente, per rispetto ai colleghi non voglio ripetere tutte le considerazioni che sono già state fatte e che condivido ma, mi soffermo solo su solo su una valutazione che credo importante. Su questi argomenti, così seri e così necessari per la sanità, maggioranza e opposizione hanno trovato un'armonia; ha fatto un ottimo lavoro il relatore, come credo abbia fatto un ottimo lavoro la Commissione, e il Ministero ha recepito diversi suggerimenti. Voglio ricordare che alcuni di quei suggerimenti sono consequenziali anche ad un'azione politica svolta nelle scorse legislature, che quindi segue un filo conduttore che porta ad una razionalizzazione della burocrazia in campo sanitario, soprattutto

inadatti e, soprattutto, non opportuni. Sicuramente questo provvedimento introduce anche qualcosa

Sapete benissimo che il sistema farmaceutico svolge in Italia un ruolo fondamentale, è parte integrante del Sistema sanitario nazionale, sicuramente è un presidio importantissimo anche nella prevenzione, perché, soprattutto nel quadro di una riduzione degli interventi di pronto soccorso, avere delle farmacie a cui rivolgersi e dove trovare personale qualificato anche nei giorni di festa è un vantaggio non indifferente. Ecco perché molti colleghi hanno presentato disegni di legge nei quali si richiedeva, ad esempio, un numero di farmacie maggiore e, quindi, un numero minore di abitanti per farmacia.

per far tesoro di una siffatta armonia su argomenti così seri che vanno al di là dello schieramento e del colore politico che tutti noi rappresentiamo

materia che richiederebbe una profonda riflessione e una competenza che, con tutto il rispetto per i colleghi della 10ª Commissione, non può interessare soltanto il campo dell'economia e delle attività produttive, ma deve riguardare soprattutto la sanità

anche a normative già presenti nel decreto. Inoltre, ricordo che è istituito presso il Ministero un tavolo di concertazione con i pubblici esercizi per la riduzione dell'uso dell'alcol e credo che queste norme, che interessano le modalità di vendita, vadano ulteriormente concordate. Su questi emendamenti,

l'incrocio dei dati tra pubbliche amministrazioni, vale a dire tra ASL e amministrazioni scolastiche, rispetto alle certificazioni sia molto più efficace dell'autocertificazione così come è oggi prevista:

Il Governo esprime grande soddisfazione per l'approvazione del provvedimento e ringrazia il relatore e la Commissione

Passiamo alla votazione

fare attenzione alla semplificazione anche della certificazione, ossia che in qualche modo venga data una possibilità di certificazione molto facile per il trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza. Ciò significa che avremmo in qualche modo l'apertura di un mercato o quanto meno un possibile abuso da parte delle tossicodipendenze

il cui testo

vuole favorire le terapie domiciliari per il dolore severo di qualunque natura, ma concederle anche a chi sfortunatamente deve fare una terapia sostitutiva e non può muoversi dal domicilio. È responsabilità del medico che prescrive accertare se il paziente può o meno muoversi dal domicilio; non credo che dobbiamo punire queste persone.

estremamente più severe, che possono anche arrivare a una piccola modifica del codice della strada. Pertanto, riteniamo che l'approvazione dell'emendamento 9.0.200 possa essere collegato all'approvazione

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della Lega Nord al provvedimento

a nome dei Gruppi della Sinistra-L'Arcobaleno - e non lo faccio per iscritto visto che non siamo intervenuti nella discussione generale - perché credo vada realmente sottolineata l'importanza di questo provvedimento

Vorrei citare alcuni elementi che abbiamo eliminato oggi, oltre al certificato di sana e robusta costituzione fisica per l'iscrizione a corsi ed a concorsi

l'evidenza scientifica in questo momento e soprattutto l'Istituto superiore di sanità stanno andando, così come in tutto il resto dell'Europa, verso l'eliminazione dell'obbligo vaccinale.

estremamente positiva - ha inserito una particolare attenzione alla salute dei bambini attraverso due obbligazioni: con la prima, che sicuramente dovrà essere rivista ed integrata all'interno della contrattazione collettiva con i pediatri di libera scelta, almeno una volta l'anno, il pediatra è tenuto a provvedere ad un bilancio di salute. Con la seconda, ancora più pregnante - sono molto

la piccola Eleonora, a Bari, nel quartiere Enziteto, era morta di fame. In quattro anni di vita nessun pediatra l'aveva mai visitata, in quanto i suoi genitori, per povertà materiale e relazionale, relazionale, non avevano per lei scelto un pediatra. La possibilità che lo Stato assegni il diritto alla salute ad ogni bambino al momento della nascita, indipendentemente dalle scelte dei genitori, è un momento di grande civiltà ed importanza. Altri colleghi hanno poi

per me, come membro della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, è particolarmente importante, perché prevede i registri nominativi sulle cause di morte. Oggi ci troviamo in grandi difficoltà nella nostra Commissione,

anche coloro che non sono della Commissione sanità, ad approfondirli, perché credo che nei loro collegi riceveranno da parte dei cittadini numerosi ringraziamenti al riguardo.

che sono risultati estremamente obsoleti nel corso degli anni. Un'operazione di pulizia e di semplificazione che è indirizzata ad un'eliminazione della burocrazia, spesso veramente molto pesante e che si traduce anche in una grossa perdita di tempo per le persone. Quindi, questo è il primo dato estremamente interessante che vogliamo rilevare. La seconda gamba riguarda la riorganizzazione delle competenze (chi e che cosa deve fare senza andarsi a pestare i piedi): riorganizzazione delle competenze per quel che riguarda le ASL, le Regioni e lo Stato. Finalmente anche su questo si mettono dei punti chiari e fermi. Le persone non dovranno rincorrere i diversi enti, ma potranno direttamente andare da colui che per competenza è predisposto a dare quel tipo di certificazione. La terza gamba viene rappresentata -

perché questo permette alla Regione, ma anche allo Stato di avere una fotografia perfetta di tutto il nostro territorio. Questo significa poter statisticamente capire esattamente qual è il grado di salute delle nostre Regioni e quanto incidono le patologie a livello epidemiologico sul territorio. Allo Stato e alle Regioni ciò permetterebbe di allocare molto meglio le risorse da destinare. quarta gamba riguarda la semplificazione dei farmaci contro il dolore di qualsiasi entità. Il dolore è una cosa che nessuno di noi vorrebbe provare sulla propria pelle. Siamo purtroppo gli ultimi in Europa - peggio di noi fa soltanto la Grecia - nell'uso degli oppiacei per contrastare il dolore non soltanto oncologico, ma anche quello severo. Credo, quindi, che questa semplificazione possa aiutare insieme ad una nuova

con le piante organiche avocando ancora a sé il principio che la farmacia è uno strumento di presidio sanitario sul territorio dello Stato.

Il relatore, senatore Cossutta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

Presidente, mossi da sollecitudine e da senso di solidarietà verso il Movimento della Palestina siamo giunti, su proposta del Governo, ad avallare - e stiamo di fatto avallando - un finanziamento a sostegno del Governo italiano in ordine al concorso per le spese sostenute dal Movimento della Palestina per la propria rappresentanza sul nostro territorio nazionale. La mia domanda è se questo senso di sollecitudine, questa sensibilità politica, questo senso di solidarietà

Non voglio creare intralcio, né mancare di riguardo agli impegni presi, soltanto se dico qualche parola in più rispetto a ciò che si attendeva è perché vorrei rivolgermi a quest'Aula. A meno che non mi si valuti una persona poco avveduta, capisco che il mio ordine del giorno può avere soddisfazione eventuale solo dal sostegno sensibile da parte della opposizione. Siamo in pochi della mia parte politica, eppure ci conto, perché questo ordine del giorno trascende

per le vessazioni cui è sottoposta quella popolazione e quella minoranza, soprattutto da parte del vicino Marocco. Quindi, sottopongo alla sensibilità e alla benevolenza dei colleghi della maggioranza questo ordine del giorno e altresì

da parte di Hamas, ancora oggi c'è un atteggiamento di chiusura. Pertanto, comprendendo le ragioni dello stanziamento che oggi intendiamo

ordine del giorno sostenga la Presidenza dell'Autorità nazionale palestinese, ricordando altresì che Hamas ha posto in essere comportamenti aggressivi ed omicidi nei confronti dei palestinesi che si riconoscono in Al Fatah.

anche «ad ogni altro movimento autonomista non in armi»: francamente mi sembra poco pertinente anche rispetto all'oggetto della discussione che stiamo svolgendo. Quindi, invito il proponente a ritirarlo,

L'ordine del giorno del senatore Fruscio nasce da una motivazione ben più ampia di quella poi riformulata dal senatore infatti, che una analoga richiesta sia avanzata «in favore di ogni altro movimento autonomista non in armi».

Ribadisco l'inaccettabilità per il Governo di questo ordine del giorno, perché se iniziamo ad introdurre un meccanismo di sostegno da parte del Governo a tutte le realtà autonomiste anche non in armi, come il Fronte Polisario, arriveremmo ad avere, in realtà, alcune centinaia di

Il tema è semplicemente questo. L'Autorità nazionale palestinese ha un *iter* storico, anche nell'ambito delle Nazioni unite, del tutto particolare.

Noi diciamo che la Presidenza dell'Autorità nazionale palestinese fa qualcosa con Hamas, assolutamente. Abbiamo ben presenti la grossa difficoltà e il grosso sforzo che sta compiendo la Presidenza nazionale palestinese. Semplicemente ribadiamo la solidarietà alla Presidenza nazionale palestinese, al processo di pace in essere, ed impegniamo il Governo a mantenere le cose così come stanno, cioè

per cui sono destinati e non ad altro, in particolare non vadano ad una organizzazione che ha nel suo statuto, nella sua carta fondamentale, dichiarazioni che si riferiscono alla necessità della distruzione di un Stato sovrano membro delle Nazioni Unite. Per cui francamente non riesco a votare altrimenti che a favore di questo ordine del giorno.

Allora, o chiediamo di trasformare il dono in un finanziamento e pretendiamo un rendiconto contabile di quello che diamo all'ANP, ma non c'entra niente Hamas, gli si deve chiedere il rendiconto contabile, altrimenti non è una donazione ma un'altra cosa. A parte il fatto che, comunque, nell'Autorità nazionale palestinese fino a 4‑5 mesi fa erano comprese tutte le organizzazioni politiche organizzazioni politiche e nessuno di noi può costringere l'ANP a tenere un atteggiamento diverso da quello che responsabilmente si assume da sola. Noi possiamo, qualora avessimo questo dubbio, decidere di non dare più questa donazione all'Autorità nazionale palestinese.

nazionale palestinese, ben identificata a livello internazionale e anche in ambito Nazioni Unite. Ribadisco la differenza rispetto all'ordine

in questo modo da Governi di diverso colore. Non si può fare diversamente anche in questa sede. Le considerazioni svolte dal relatore e dal collega Mantica sono totalmente condivisibili, quindi continuo a mantenere un parere contrario.

giorno reca: «Informativa urgente del Governo sui recenti attentati in Algeria». Come precedentemente comunicato, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo

esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, negli ultimi mesi si è assistito ad una preoccupante recrudescenza dell'attività dei gruppi terroristici algerini che nel corso del 2007 hanno provocato numerose vittime, sia tra i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'Esercito, che tra la popolazione civile. Tale fenomeno va inquadrato nel rifiuto che fin dall'inizio le frange più estremistiche dell'islamismo radicale hanno opposto alla politica di riconciliazione nazionale voluta dal presidente Bouteflika. Uno degli aspetti più significativi della politica attuata dal presidente Bouteflika è stato infatti il processo di normalizzazione della situazione interna dopo l'offensiva terroristica degli anni '90. Un processo realizzato anche attraverso il coinvolgimento attivo degli algerini, chiamati alle urne per l'approvazione del programma di riconciliazione nazionale proposto dal Presidente. Nel settembre 1999 un *referendum* popolare ha confermato la «legge sulla concordia civile», adottata a luglio dello stesso anno, ed il 29 settembre 2005 si è svolto il *referendum* popolare per l'approvazione della «Carta per la pace e la riconciliazione nazionale». L'obiettivo è la chiusura definitiva della pagina del terrorismo, prevedendo in particolare l'estinzione delle procedure giudiziarie a carico di coloro che hanno abbandonato ogni attività armata e si sono consegnati alle autorità (ad eccezione di quanti si sono resi responsabili di massacri collettivi, di stupri o di attentati con uso di esplosivi perpetrati in luoghi pubblici). Un consistente numero di terroristi ha sottoscritto l'amnistia proposta dal presidente Bouteflika, collaborando con le autorità algerine nella lotta contro i gruppi armati ancora attivi, nel frattempo riorganizzatisi sotto la sigla GSPC (Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento). Questo gruppo ha riunito i terroristi irriducibili ed è ritenuto responsabile di molte stragi di civili algerini avvenute negli ultimi anni, anche dell'azione che vide il rapimento nel 2003 di diciassette turisti europei, liberati in un *blitz* delle forze speciali algerine dopo tre mesi di prigionia. Alla fine del 2006 il GSPC ha annunciato di aver aderito alla rete di Al Qaeda, modificando la propria denominazione in Organizzazione di Al Qaeda per i Paesi del Maghreb, come confermato l'11 settembre scorso da Ayman al Ayman al Zawahiri, braccio destro di Osama Bin Laden. Alla nuova sigla terroristica sono stati attribuiti i drammatici attentati compiuti in Algeria nel corso del 2007, tra cui, oltre alle esplosioni di ieri, vanno ricordati i seguenti: 11 aprile, due autobombe esplodono ad Algeri provocando la morte di 33 persone e oltre 200 feriti; 11 luglio, un *kamikaze* al volante di un'autobomba si fa esplodere presso una caserma nella regione della Kabilia uccidendo otto persone; 6 settembre, un attentato suicida causa 20 morti e 107 feriti a Batna, poco prima dell'arrivo del presidente Bouteflika; 8 settembre, un'autobomba esplode presso gli alloggi della guardia costiera nel porto di Dellys e provoca la morte di 37 persone. Del recente deterioramento delle condizioni di sicurezza in Algeria sono state fornite notizie e particolari sul sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it, nel quale si consiglia ai connazionali presenti nel Paese di adottare un atteggiamento di cautela in ragione del rischio terroristico, suscettibile di colpire anche interessi occidentali. L'Unità di crisi della Farnesina e l'Ambasciata ad Algeri hanno inoltre provveduto a sensibilizzare, attraverso periodiche riunioni informative, i responsabili delle imprese italiane operanti *in loco*. L'attentato che ha colpito Algeri nella mattinata dell'11 dicembre ha preso di mira le sedi del Consiglio costituzionale (recentemente inaugurata, attigua alla Corte suprema e ad un centro commerciale) e delle Nazioni Unite, entrambe situate in due quartieri residenziali in cui hanno sede rappresentanze diplomatiche e società straniere. Non appena appreso del duplice attentato, l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri, in collegamento con l'Ambasciata ad Algeri, ha verificato l'eventuale coinvolgimento di connazionali, attraverso controlli nelle banche dati, contatti telefonici con le imprese italiane presenti in Algeria e verifiche dirette presso gli ospedali dove sono stati trasportati i numerosi feriti. A seguito di tali riscontri è stato possibile confermare che nessun italiano è rimasto coinvolto nelle esplosioni. I dati non definitivi del duplice attentato di ieri, rivendicato con un comunicato diffuso su Internet dall'organizzazione Al Qaeda per i Paesi del Maghreb, parlano di almeno 26 morti e 177 feriti, molti dei quali studenti universitari di età compresa fra i 18 e i 25 anni, alcuni bambini e numerosi funzionari dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale, l'Algeria è particolarmente attiva sia a livello multilaterale che bilaterale. In particolare, si segnala che ad Algeri ha sede il CAERT (Centro di ricerche e studi antiterrorismo istituito dall'Unione africana nell'ottobre 2004), che svolge un'importante attività di coordinamento regionale nella lotta al terrorismo ed in favore del quale sia la Commissione Europea che, in maniera indipendente, l'Italia hanno previsto per quest'anno dei contributi *ad hoc*. Si segnala altresì che l'Algeria ha recentemente preso parte all'iniziativa della NATO per la lotta contro il terrorismo denominata *Active Endeavour*. l'Algeria è per l'Italia un *partner* di primaria importanza, in particolare nel contesto della strategia intesa a rilanciare la vocazione mediterranea della politica estera italiana. Testimonianza significativa del ruolo centrale dell'Algeria è stato il vertice italo-algerino, il primo del suo genere con un *partner* della sponda Sud del Mediterraneo, tenuto ad Alghero il 14 novembre scorso. Anche per questo, oltre che nel quadro più generale delle iniziative internazionali di contrasto al terrorismo, l'Italia collabora strettamente con l'Algeria sul piano bilaterale ed ha firmato nel 1999 uno specifico accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione illegale, già ratificato dall'Italia ed in via di ratifica da parte algerina. c'è dunque una grande preoccupazione, moltiplicata dall'attentato di questa mattina a Beirut: come noto, è stato assassinato il vice comandante delle Forze armate libanesi proprio mentre il comandante delle Forze armate libanesi appare essere il candidato più probabile per l'elezione a Presidente della Repubblica. La preoccupazione è accresciuta dal fatto che l'attentato di Algeri è rivolto anche contro le Nazioni Unite sotto la cui bandiera stanno i nostri soldati in Libano.

di ieri il secondo attentato in Algeria dopo quello avvenuto l'11 aprile scorso che ha causato 33 morti e 300 feriti. Si tratta di una strage che ancora non vede una rivendicazione certa, ma che è riconducibile alla mano insanguinata di Al Qaeda, non tanto perché il numero 11, scelto dagli attentatori, rappresenti qualcosa nella simbologia dell'Islam, quanto perché, dopo Ground Zero, l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, l'11 di ogni mese è diventato come una firma, un segno di assoluta riconoscibilità, un guanto di sfida contro l'Occidente e contro i «crociati», per utilizzare un termine caro alla Jihad, in un'ottica di guerra santa dei figli di Maometto al Male-Occidente. Come mai, dunque, rivendicare la strage di ieri di Algeri, che ha provocato una trentina di morti, fra cui cinque stranieri, e ventotto feriti? Si tratta quasi certamente di una riflessione che il "qaedismo" ha fatto rispetto alla guerra globale e alla necessità di riprendere un'offensiva integralista che parta proprio dal Governo algerino per condurre altrove. In Algeria, infatti, dopo il sangue versato e gli scontri (circa 150.000 morti, soprattutto fra giovani e bambini), è prevalsa la linea che impedisce una sovrapposizione tra religione e Stato, fatto assai raro per la cultura islamica. Ad oggi, però, dopo l'intervento di pace della Coalizione dei volenterosi in Iraq, che ha fatto raffreddare i bollenti spiriti antiamericani, nonostante vi siano sacche di terrorismo e di ribelli ancora in azione, è proprio in Algeria (dove il Governo non è in mano agli integralisti) che il terrorismo può trovare terreno fecondo, anche facendo leva sui problemi socio-economici che questo Stato presenta, fra cui un numero molto alto di disoccupati di età inferiore ai 30 anni. Voglio ricordare a tutti noi che l'Algeria è un Paese chiave per il Mediterraneo Orientale ed in modo particolare per il nostro Paese, che ha da sempre fitti scambi economici importanti, soprattutto per quanto concerne l'approvvigionamento energetico, fattore che ha contribuito a fare dell'Algeria lo Stato, fra i Paesi del Medio Oriente, con il PIL più alto. Tra l'altro, sono in corso progetti di costruzione di oleodotti ed è dunque scontato

sono in corso progetti di costruzione di oleodotti ed è dunque scontato che l'Italia debba continuare ad avere rapporti continuativi e frequenti con l'Algeria.

per provare ad offrire uno sbocco, una via d'uscita da quella che può rivelarsi una polveriera a due passi dall'Europa e ad un soffio dal nostro territorio, con tutte le ripercussioni che questo avrebbe, sia per l'accaparramento delle risorse energetiche che per gli scambi economici più in generale. Mai come ora il Governo algerino è in difficoltà, subisce la pressione di questi gruppi terroristi che vorrebbero imporre la Sharjah. Proprio perché in Algeria vige il divieto per i partiti politici di richiamarsi alla religione, si dimostra che il vero argine all'islamismo terrorista sono le stesse società musulmane. Questa riflessione deve essere accompagnata da un'altra, che urge fare con un certo rigore, relativa all'immigrazione. Il fenomeno migratorio è vasto e complesso e non si può certo pretendere di risolverlo con un tratto di penna o con uno *speech*. Il problema però è serio, perché riguarda anche la sicurezza del nostro Paese. Anche in questo campo cosa intende fare il Governo? Questa è la domanda che noi le poniamo, signor vice ministro. Vuole proseguire con la politica delle frontiere aperte a tutti in modo indistinto, tanto cara al ministro Ferrero, oppure intende procedere in modo meno permissivo e più europeo, come ha più volte sollecitato il commissario Frattini? Non è un dettaglio, questo: i cittadini, che subiscono quest'angoscia e questo senso di vulnerabilità permanente che la guerra asimmetrica induce (ciascuno di noi può essere colpito in qualsiasi momento),

all'immigrazione clandestina e alla predicazione degli Imam in odore di terrorismo. Con queste considerazioni, signor Vice ministro, intendiamo sollecitare il Governo ad assumere tutte quelle iniziative di chiarezza, affinché - come ricordava anche lei, nella sua relazione - si possa definire meglio una strategia dell'Italia, non solo nel quadro europeo, ma anche nella politica del Medio Oriente.

un massacro collettivo (com'è stato detto dal Governo molto correttamente), di un atto barbarico, con vittime civili, giovani, anche bambini, studenti. Oltre al cordoglio che dobbiamo esprimere al Governo, al popolo, alle famiglie credo dobbiamo sottolineare che queste azioni, tipiche del "qaedismo", sono svolte per seminare terrore,

è il giorno 11: è la firma, il marchio dall'11 settembre del 2001, alle Torri gemelle, al Pentagono e anche in Algeria

e poi all'11 dicembre, appunto, all'Agenzia per lo sviluppo delle Nazioni Unite e al Commissariato per i rifugiati. È stata colpita, ancora una volta, l'organizzazione delle Nazioni Unite, come a Baghdad, in quel tragico 19 agosto 2003, quando fu distrutta la sede dell'ONU e trovò la morte il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite, Sergio Vieira de Mello. Questa, come le precedenti, è una barbara azione, basata su una guerra ideologica jihadista,

sembra che siano stati richiamati terroristi che hanno operato in Iraq e che anche il Gruppo salafita confluisca e dia supporto operativo all'organizzazione di Osama bin Laden. Allora, è necessario, fortemente necessario, che la comunità internazionale controbatta efficacemente queste azioni, che controbatta con l'informazione ma, soprattutto, promuovendo lo sviluppo economico e sociale. Laddove non c'è la capacità e l'esistenza di una tendenza allo sviluppo economico e sociale, là può attecchire il terrorismo. Altrimenti, la propaganda e l'azione di Al Qaeda fanno proseliti, imponendo con il terrore il suo potere.

dal 1992, la violenza terroristica ha causato oltre 200.000 morti. Esistono però anche altri motivi di contrapposizione interna ai gruppi qaedisti. Il gruppo duro e spietata di Abdelmalek Droukal avrebbe addirittura organizzato questo orrendo attentato - che, come ho detto, non risparmia i civili - anche per ragioni di potere interno, interno, di supremazia nell'ambito delle stesse organizzazioni terroristiche: direi, assurdamente, per acquisire meriti nei confronti di Al Zawahiri.

La stessa Unione Europea deve esprimere ancora maggiore attenzione nei confronti di una realtà geografica che è alle nostre porte e deve quindi operare con ancora più determinazione e impegno. L'Unione Europea si appresta ad approvare il Trattato di Lisbona,

si deve inviare un segno concreto, un segno operativo per agire con ancora più intensità, con più mezzi e più determinazione in questa area e, soprattutto, in Algeria. in Algeria. Da questo punto di vista, il Governo italiano, dopo aver evidenziato, come ha fatto il Governo, gli accordi di collaborazione contro il terrorismo

iniziative dell'intera Unione Europea. Infatti, questa deve essere la vocazione e la grande capacità di questa nostra area per poter fare in modo che in un'area così limitrofa non s'inneschi questo processo

non ci ha comunicato grandi novità anche perché, leggendo la stampa internazionale, già oggi un quotidiano del Cairo, Al Ahram, ha parlato della rivendicazione da parte Al Qaeda del Maghreb islamico della responsabilità degli attentati di ieri. Poteva sembrare anche superfluo in quanto questa ripetizione della data dell'11 del mese sembra ormai un sigillo utilizzato per marchiare, quasi come la stella a cinque punte degli anni di piombo, che ha caratterizzato appunto gli anni bui della storia di questo Paese. Una cosa in più abbiamo scoperto leggendo sempre la stampa internazionale: la sede della Corte suprema di Algeri casualmente si trova in una viuzza che si chiama proprio «Via dell'11 dicembre».

ha dovuto ammettere una "responsabilità amministrativa" e ha detto che la loro colpa è stata quella di aver abbassato la guardia. Nei confronti di questa grande organizzazione invisibile nessuno Stato islamico, men che meno occidentale, può permettersi il lusso di abbassare la guardia. Se guardiamo cosa sta accadendo in questo momento storico in Italia, vi è un Governo che non ha politiche. Non ha politiche economiche,

sulle scelte previdenziali si rischieranno spaccature di maggioranza; il guaio è che non ci sono politiche comuni della sicurezza in in questa maggioranza. D'altronde, con visioni così difformi del mondo, una compagine così mal assortita, non può prendere decisioni lineari e serie. Vi sono due modi di vivere gli eventi, di guardare con la lente il mondo. Il peggio è successo a questo Paese, all'Italia: ha messo insieme ciò che era inconciliabile. Veniamo al punto: non ci resta che appellarci a forme di governo territoriali, apparentemente meno efficaci, ma che a questo punto garantiscono molto di più.

l'arrivo di tutte quelle persone che non dimostrano di essere qua con un ruolo, di avere un lavoro, *ergo* un reddito, *ergo* di potersi mantenere,

Dal 2001 il terrorismo internazionale è stato il nemico invisibile del mondo occidentale: ha pagato forse il prezzo più alto l'America, ma anche Madrid, la Spagna non è stata immune. Londra ha pianto altrettanto i propri morti. In Medio Oriente non sappiamo più come definirlo, nel senso che ormai probabilmente non è nemmeno più controllabile il fenomeno: il Libano piange oggi quello che poteva essere probabilmente un futuro *premier*; Israele ogni altro giorno deve piangere morti e si deve difendere investendo il 40 per cento del proprio bilancio in sicurezza: non vi è Stato al mondo che deve fare questi sforzi. Oggi, l'Algeria: guardate che sono

l'uccisione di un consigliere politico di Al Qaeda, un esponente algerino, ucciso tempo fa dalle forze di sicurezza algerine.

che questo fenomeno, l'Islam fondamentalista, riesca a dare un timbro e probabilmente persuadere, anche le formazioni non estremiste, o con

È questo l'Islam con il quale noi continuiamo a dire che ci dovremmo confrontare, perché sarà quello che dominerà nei Paesi in cui riuscirà a schiacciare la parte dialogante, la parte più debole, cioè la parte

finiremo per dare l'idea che anche in Europa si potrà continuare a diffondere quel tipo di ragionamento con quel tipo di metodo violento. L'invito che vorremmo rivolgere al Ministro ed a tutto il Governo è di mettere in atto tutte le misure e tutte le politiche che offrano la maggior sicurezza per i nostri cittadini e per tutto il nostro Paese.

del vice ministro Intini, che ha dato conto delle cose successe e ha posto in essere anche alcuni atti importanti dal punto di vista dell'iniziativa politica. È chiaro che in questo discorso rientra, in primo luogo, la condanna degli attentati, il cordoglio per i morti, per la crudeltà e l'efferatezza dei fatti di questi giorni, efferatezza e crudeltà che spesso abbiamo visto negli attentati in Algeria. Siamo stati avvezzi a sentire notizie anche ben più pesanti. la condanna si accompagna alla solidarietà con le persone e le istituzioni colpite, con la Corte suprema algerina (cui la nostra Corte costituzionale ha inviato giustamente un telegramma di solidarietà molto importante). È questo un punto di grande riflessione. Ora però questi attentati, che seguono ad altri attentati, come ha ricordato il vice ministro Intini e come abbiamo letto in questi giorni sui giornali

che tali attentati producono un accrescimento del terrorismo; cioè, non vi è sosta negli attacchi terroristici.

tanti morti e tanti *kamikaze*. I *kamikaze* sono ragazzi, talvolta di quattordici anni. La polizia continua a scoprire adolescenti implicati in azioni terroristiche. C'è qualcosa di inquietante in queste parole e in questi fatti. L'Algeria è nello stesso tempo anche il Paese che ha il maggior sviluppo economico in Africa dopo il Sudafrica; pur tuttavia, ciò che sembrava risolto, oggi sembra di nuovo attaccato, se non compromesso.

anzi lo hanno allargato. Il fronte mediterraneo - come qui è stato ricordato - è quello su cui maggiormente questi attacchi si allargano. Quindi, c'è un impegno importante. Devo dire al senatore Divina - che ora non vedo - che la maggiore sicurezza non dipende dai sindaci del Nord-Est (che peraltro, secondo me, vanno contro la legge),

se in questi anni di guerra questo fronte si è allargato; c'è oggi bisogno di costruire una nuova svolta d'iniziativa politica. La guerra civile in Algeria è costata più di 150.000 morti, qualcuno dice 200.000. Pensavamo che aver soffocato la parte estremista avesse risolto il problema, ma ciò non è

Allora, penso che su questo punto c'è una riflessione che va oltre e che non può essere esaurita in questa discussione perché - ringrazio molto, peraltro, il Vice ministro perché ci ha dato alcune utili indicazioni - c'è bisogno di una svolta vera. una svolta vera. Il clima di guerra così forte in tutto il Medio Oriente non può continuare all'infinito:

colpito. Mi pare che questo punto di vista, però, rischia di essere appannato e noi in questo Paese non dobbiamo farlo appannare:

La sicurezza dipende da questo accrescimento della politica di pace, cioè dal fatto che la stessa politica estera dell'Europa sia costruita su questo. Penso che da questo

formulato ieri in quest'Aula dopo i tragici fatti di Algeri. Credo che esprimere solidarietà al popolo algerino sia un fatto scontato. Ritengo che, come al solito, quando avvengono questi fatti, al di là dell'emozione del momento, occorra fare qualche riflessione e soprattutto capire come si possa esprimere sul sul piano politico e sul piano dei rapporti bilaterali una vera solidarietà del popolo e del Governo italiano all'Algeria. Devo innanzitutto dire a chi è intervenuto prima di me che equiparare la situazione algerina ad altre situazioni in Medio Oriente non è corretto: l'Algeria vive da più di quindici anni una vicenda drammatica di guerra civile e di esplosione del terrorismo islamico e l'Algeria - va riconosciuto è da quindici anni il fronte primo in cui anche l'Europa combatte la sua battaglia contro il terrorismo. L'Algeria vive una vicenda legata ad una scelta per certi versi non democratica, quando molti anni fa furono annullate le elezioni che avevano visto la vittoria del FIS (Fronte islamico di salvezza), da cui ebbe poi origine la grande tragedia della guerra civile algerina. la situazione dell'Algeria per quello che è; credo che alcuni aiuti si possano dare, politicamente e concretamente. è un Paese nel quale esiste una centrale per la lotta al terrorismo per tutto il Continente africano cui l'Italia collabora; credo sia questo il momento di rafforzare la nostra collaborazione e il nostro impegno nei confronti di uno strumento che l'Algeria si è data e che certamente può servire anche a noi per meglio gestire le vicende che riguardano complessivamente il Mediterraneo. L'Algeria ha bisogno, secondo noi, e va aiutata nella costruzione vera, reale e concreta dell'Unione del Maghreb Arabo, perché questa grande area (che occuperebbe Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia) potrebbe diventare l'interlocutore privilegiato dell'Europa e probabilmente una frontiera vera, reale nella battaglia al terrorismo. Aiutare l'UMA, la costruzione di questa realtà che resta sulla carta da molti anni significa, per esempio, signor Ministro, avere da parte del Governo italiano

Marocco; non dobbiamo infatti dimenticare che, mentre parliamo di Unione del Maghreb Arabo, la frontiera tra il Marocco e l'Algeria è interrotta da più di vent'anni.

che su questo piano manca molto, viste le posizioni differenziate di Spagna e di Francia. Quando invochiamo una politica estera europea, senza fare discorsi di grandissimo livello (esiste un problema concreto che interessa l'Europa, un problema di stabilizzazione Esiste il problema di un processo di Barcellona che ha compiuto più di dieci anni (credo vada ormai per i dodici anni), che non funziona e non si sviluppa. Il processo di Barcellona significava e significa creare un grande mercato, nel Mediterraneo, di scambio di merci e di persone, cioè avviare un processo innovativo e diverso rispetto ai sistemi attuali; significa associare questi Paesi alla realtà dell'Unione Europea. Anche in questo caso, credo che l'Europa debba assumersi le proprie doverose responsabilità, rivolgendole doverose responsabilità, rivolgendole al mondo del Nord Africa; i processi di democrazia in Algeria e Tunisia sono sostanzialmente bloccati, anche se alcune forme di democrazia, come le elezioni, certamente vanno riscontrate, come è fermo il processo democratico

di un rapporto bilaterale più stretto che a mio giudizio va al di là dell'interesse economico. Esiste la possibilità di un rafforzamento della cooperazione sul piano politico. Voglio ricordare che l'Algeria si è trovata spesso al fianco dell'Italia, ad esempio, su questioni come la riforma del Consiglio di Sicurezza o la riforma dell'ONU. Esistono possibilità di incrementare e implementare i nostri rapporti sul piano culturale, più volte: anche recentemente abbiamo approvato la ratifica di un accordo con l'Algeria in materia di produzione culturale. Voglio ricordare le richieste che più volte l'Algeria ha indirizzato all'Italia per la conservazione del suo più grande museo all'aperto nella zona del Tassili. zona del Tassili. Esistono possibilità concrete, al di là di una manifestazione di solidarietà, per far capire quanto sia importante per l'Italia, per la sua politica estera e per il suo ruolo nel Mediterraneo, un rapporto - oserei dire - privilegiato con l'Algeria.

che dovrebbe far riflettere molto coloro che pensano che lo sviluppo del terrorismo islamico sia strettamente legato all'operazione - peggio ancora - alla missione *Enduring Freedom* in Afghanistan. Evidentemente, è un processo molto più complicato: l'Algeria non ha mai subito, dalla sua indipendenza ad oggi, occupazioni straniere, e non ci sono attualmente presenze militari straniere;

partecipazione dei cittadini al Governo del Paese. Credo che questa sia un grande responsabilità dell'Europa e stia soprattutto nella capacità dell'Europa operare a fianco delle forze islamiche moderate e democratiche, riconoscendo il valore della dissidenza - laddove esiste ed è presente in molti Paesi - e, soprattutto, premendo perché l'evoluzione della democrazia in quei Paesi non si blocchi

che vede i figli dei *leader* assumere ruoli primari nell'ambito dello sviluppo del Paese. Ritengo, signor Vice Ministro, che il Governo italiano dovrebbe riprendere un'iniziativa più forte. più forte. Manifestare solidarietà assume un significato nel momento della forte emozione di fronte ai cadaveri di Algeri, ma credo che l'Italia all'Algeria debba qualcosa di molto più importante.

Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la sua relazione così puntuale.

si associno agli atti di condanna che il Governo ha saputo esprimere ad una Nazione a noi così vicina. Occorrono

i telegiornali di ieri, che hanno dato la notizia dell'attentato di Algeri non in prima, ma in seconda, terza o quarta battuta, come se si fosse di un evento minore. Questo, invece, è un tragico evento di grandissima portata, che segue un intensificarsi dell'azione terroristica in Algeria, che negli ultimi due anni si è fatta estremamente intensa.

nei quali potrebbero avvenire atti terroristici. Cosa posso dire di più di quanto detto molto bene da altri colleghi,

e ai Paesi del Maghreb. In Francia, in Spagna e in Italia la maggioranza degli immigrati proviene dal Maghreb: anche se non in particolare dall'Algeria, dalla grande area del Maghreb. Siamo quindi umanamente, socialmente legati a questa realtà nordafricana e non possiamo invocare

grandi comunità maghrebine che i nostri Paesi ospitano. Questo ci deve incitare a porre in essere quella maggiore cooperazione con questi Paesi invocata da vari colleghi che hanno preso la parola.

consumiamo probabilmente un gas che proviene dall'Algeria. Il nuovo gasdotto, pianificato e approvato nel vertice di Alghero, unirà Algeri con la Sardegna e la Sardegna con la Penisola. I contratti di fornitura di metano e di energia sono stati prorogati fino al 2019. Quindi noi dipendiamo e siamo fortemente connessi politicamente ed economicamente con questo Paese. 150 o 200 imprese grandi e medio-grandi lavorano in Algeria. Ci sono programmi per 60 miliardi di euro di lavori pubblici,

Il senatore Mantica ha citato, per esempio, il piano culturale, il piano dell'insegnamento, della cooperazione universitaria, della cooperazione culturale, fatto importantissimo. Troppo lontani sono ancora i Paesi del Maghreb dalla psicologia italiana; un avvicinamento può essere fatto e il Governo può aiutare in questo. Occorre, Occorre, naturalmente, cooperazione nell' ambito del contrasto al terrorismo. È stata citata la centrale che già esiste in Algeria per l'Africa, cui collabora collabora l'Italia; credo vada rafforzata questa cooperazione e penso anche che la politica migratoria non abbia nulla a che fare con il contrasto al terrorismo. Ricordiamo che 23 dei 24 attentatori delle Torri gemelle erano legalmente residenti, o legalmente entrati, negli Stati Uniti; ricordiamo che gli attentatori di Londra erano cittadini britannici. Il contrasto al terrorismo non si fa chiudendo le porte all'immigrazione, ma rafforzando l'*intelligence*. Vorrei anche puntualizzare, rispetto a quanto ha sostenuto il senatore Baccini, che l'Italia non persegue una politica di porte aperte; l'Italia sta proseguendo

Quindi, forte cooperazione in ambito economico, forte cooperazione in ambito mediterraneo. Giustamente è stato evocato il processo di Barcellona, che troppi intoppi e rallentamenti ha avuto

del Maghreb), ci si debba anche ricordare che le nostre politiche comunitarie spesso sono in antitesi con la nostra volontà di cooperazione. Vorrei solo rammentare le politiche agricole

Non mi voglio dilungare oltre. Le notizie sono tragiche; vorrei che l'opinione pubblica italiana fosse meglio informata di ciò che avviene nel resto del bacino del Mediterraneo, essendo molto distratta sotto questo profilo. profilo. Credo che il Governo possa fare molto per rafforzare la cognizione che viviamo intorno ad un mare comune, in un mondo sempre più globalizzato, con sempre maggiori scambi culturali, umani, politici, economici questi scambi vanno mantenuti sui retti binari, anche se non è facile. Ringrazio ancora il Governo e spero prosegua secondo le linee tracciate finora, rafforzando

Grazie